comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale"***

Signora Presidente, sul tema della risoluzione che già da ieri mattina abbiamo iniziato a trattare in quest'Aula il nostro Governo, ovviamente, ha avuto modo di esprimersi in molte occasioni negli ultimi tempi, visti i fatti e gli accadimenti, e ancor più ha avuto modo di agire (anzi, ha dovuto), a mio giudizio molto bene, sia per quanto riguarda la fase delle criticità dettate dall'emergenza sia per quanto riguarda la formulazione di una politica più attenta al medio e lungo periodo.

focale della risoluzione, almeno secondo la mia interpretazione, è riassumibile nelle parole: «L'Europa deve essere più responsabile; l'Europa deve essere più Europa». Mi sembra che tale concetto, oltre ad essere fin da subito denunciato dal ministro Maroni, sia stato espresso in modo trasversale anche nel corso della discussione

possiamo andare a curare una situazione di emergenza come quella che oggi purtroppo viviamo, ma possiamo anche riuscire a prevenire ogni emergenza.

dobbiamo essere Europa nel bene, ma anche nel male, con onori e con oneri. Tuttavia, come ho detto prima, mentre l'Italia ha già dimostrato di saper fare Europa, ora deve essere l'Europa a dimostrare nei nostri confronti di essere tale. effetti, un conto è il ruolo primario quale Paese che offre la prima assistenza, un conto però è, come sta accadendo, essere lasciati soli dall'Europa.

Proprio per questo motivo, mi corre l'obbligo di ricordare l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fissa un chiaro principio di solidarietà e di equa ripartizione di responsabilità tra gli Stati membri, e questo anche sul piano finanziario,

Commissione le problematiche riguardanti l'asilo politico, che potrebbero riassumersi nel seguente quesito: spetta solo a noi, o spetta all'Europa, dividere l'onere dell'arrivo nel nostro Stato di profughi richiedenti asilo e non rimpatriabili? È una domanda che ci stiamo facendo tutti ed è una domanda, ovviamente, retorica. europea - che ho appena citato - e, ancor di più, la direttiva n. 55 del 2001 danno con chiarezza la risposta al quesito, affermando che l'Europa dovrebbe essere il primo attore in questi casi. Purtroppo l'atteggiamento europeo è andato, sta andando e continua ad andare in un'altra direzione. la commissaria dell'Unione europea agli affari interni, Cecilia Malmstrom, spiegando, ai tempi dell'immigrazione tunisina, che la procedura della direttiva n. 55 del 2001 non si può far scattare perché non c'è un flusso abbastanza rilevante di profughi. Quindi, per l'Europa sono troppo pochi gli sbarchi in Italia. Questo francamente è qualcosa che ci sentiamo non solo di criticare, ma è l'evidenza che va a criticare una dichiarazione di questo tipo. L'Italia può essere un ponte fra il Nord Africa e l'Europa, ma non per l'immigrazione verso l'Europa: l'Italia può essere un ponte tra il Nord Africa e l'Europa per la concretizzazione delle politiche comunitarie,

certo essere considerata quel lembo di terra tra confine europeo e nordafricano chiamato terra di nessuno; non può essere una sorta di bacino di contenimento predisposto a salvare l'Unione da situazioni di crisi migratoria. L'Italia o è riconosciuta dall'Europa come parte di se stessa o non lo è, ma allora lo si dica.

e in questa risoluzione, giustamente, si invita la Commissione europea a valutare la possibilità di attuare questa direttiva: una richiesta, come tutti sappiamo, già avanzata tantissime volte dal nostro Governo, particolarmente per voce del ministro Maroni, ma che non ha trovato fino ad ora alcun accoglimento da parte del *partner* europeo. Eppure, di fronte all'ondata migratoria proveniente ora dalla Libia non ci si può più trincerare, come si è fatto in passato per le ondate provenienti dalla Tunisia, dietro l'inapplicabilità di questo strumento. tale strumento è stato proprio concepito per attivare il meccanismo di solidarietà di fronte all'emergenza di un flusso importante di sfollati.

anzi, è una presa in giro. E, non a caso, l'operato del nostro ministro Maroni è stato più volte elogiato dal Capo dello Stato, che ha dichiarato testualmente di apprezzare e condividere la linea rispetto alla politica dei flussi migratori che si stanno riversando riversando sulle nostre coste in seguito alla crisi libica. In sostanza, spero che da questa nostra discussione, come già accaduto in Commissione, emerga - e vorrei rubare le parole al collega Marcenaro - la necessità di un ripensamento sull'attuale sistema europeo che assegna il compito primario di prestare aiuti umanitari allo Stato di prima accoglienza,

Infine, vanno condivise tutte le valutazioni e le proposte contenute nella risoluzione presentata dall'onorevole Provera e approvata dal Parlamento europeo il 5 aprile di quest'anno sui flussi migratori causati dall'instabilità. Pur apprezzando gli sforzi compiuti dalla Commissione europea nella recente comunicazione sulla migrazione del 4 maggio, riteniamo che siano presenti ancora delle carenze. In particolare, riteniamo che debba essere assegnato un ruolo più attivo a FRONTEX che, da strumento di semplice coordinamento, deve divenire divenire un organo operativo in grado di gestire in modo condiviso i problemi crescenti che si presentano sulle frontiere esterne dell'Unione, sulla base di quanto previsto al quinto punto delle conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni dell'11 aprile. Qui attendiamo risposte urgenti e concrete: nessun'altra presa in giro sull'impegno assunto dai Ministri. FRONTEX deve rafforzare la propria attività e avviare da subito negoziati con i Paesi rivieraschi per organizzare pattugliamenti congiunti, quindi finalmente essere Europa, nel bene e nel male. Signora Presidente, vorrei fare un'osservazione introduttiva. È vero che l'Europa ha spostato il suo baricentro di attenzione verso Nord ed Est; è vero che ha trascurato e messo all'angolo la Turchia; è vero che il processo di Barcellona si è impantanato che l'Unione Mediterranea è morta, anche se il funerale non è stato fatto: mi sono preso la briga di andare a vedere il sito dell'Unione Mediterranea ed è praticamente morto anche quello. l'Europa paga una disattenzione verso un'area del mondo vicino a noi fatta di 200 milioni di abitanti (tutto il Nord Africa)

Speriamo che le orecchie della baronessa Ashton siano ben aperte. Purtroppo, vedo già che l'attenzione dei *media* e dell'opinione pubblica europea si sta di nuovo spostando verso altre direzioni. Notavo ieri che nel nostro maggiore quotidiano nazionale

Il Trattato di Lisbona naturalmente continua a prevedere che i criteri di ammissione dei migranti all'Europa siano il dominio di ciascuno dei 27 Stati; nessuno dei 27 Stati vuole e ha mai voluto cedere una frazione di sovranità sotto questo profilo. Quindi una politica migratoria europea, per uno spazio europeo, per un mercato aperto aperto dove anche il lavoro circoli normalmente e liberamente, non esiste. Questo è il grande limite della nostra Europa.

Schengen garantiscono la perfetta mobilità. Non ci sono più i dazi, le cinte daziarie che c'erano intorno alle città. Pensate se fossero reintrodotte, se domani la Regione Toscana stabilisse, essendo in un momento difficile, di mettere le guardie ai valichi appenninici per vedere chi entra e chi esce. Per fortuna questo non accade: c'è Schengen. Questo Accordo però in qualche modo è messo in discussione. Qui è stato messo in discussione in maniera estremamente goffa per l'afflusso di migranti dalla Tunisia. Ricordiamo che questo afflusso è stato molto particolare, in un periodo estremamente particolare. Ricordo anche - tra parentesi la Tunisia ha ricevuto 360.000 rifugiati dalla Libia nel giro di due mesi (sono dati dell'UNHCR), cioè 15 volte il numero dei rifugiati in Italia dalla Tunisia, che la Tunisia ha un sesto della popolazione italiana e ha un cinquantesimo del reddito nazionale italiano, tanto per mettere le cose nelle dovute proporzioni. Effettivamente in Tunisia c'è stata un'emergenza politica che andava in qualche modo sostenuta. Ebbene, noi abbiamo dato finalmente - credo che si sia fatto bene - il permesso di sei mesi

Da qui è sorta la nota controversia con la Francia, che è stata poi risolta magicamente con l'incontro Berlusconi-Sarkozy, nel quale Berlusconi ha dato chiaramente ragione alla Francia, perché così si dice. Nella Nella lettera mandata da Van Rompuy a Barroso, infatti, si chiede la possibilità di ristabilire temporaneamente controlli alle frontiere interne in caso di difficoltà eccezionali nella gestione delle frontiere esterne comuni, si chiede all'Unione europea di convalidare l'operato del Ministro dell'interno francese, quello contro cui avevamo

non ha tenuto il punto, anzi ha fatto un voltafaccia assolutamente clamoroso. Quindi, c'è un paradosso Schengen. Nella riunione del 4 maggio, la commissaria europea Malmstrom e la Commissione si sono in qualche modo

un aumento del sostegno al partenariato e alla cooperazione con i Paesi di origine dei migranti; non si chiede una revisione di Schengen, perché questa implicherebbe un nuovo Trattato, e ciò sarebbe estremamente macchinoso e difficile, ma si chiede di reinterpretare alcune clausole di Schengen e, ancora, si propone il potenziamento di FRONTEX. Benissimo, il potenziamento di FRONTEX è nei programmi da tempo, ma anche qui c'è un nodo politico: FRONTEX deve diventare un'agenzia autonoma che fa autonomamente un certo lavoro? E politicamente a chi risponde? Risponde ai singoli Governi che lo compongono, o deve rispondere politicamente al Parlamento europeo? Questi sono grossi nodi che devono essere risolti e che non possono essere essere consegnati a delle mere dichiarazioni di principio. Questo è un problema: cosa fare di Schengen, come minimizzare la possibilità di accendere e spegnere la libera circolazione pigiando un interruttore. Questo è un problema estremamente grave: Schengen è una grande conquista, quindi ogni limitazione alla libera circolazione deve essere dettata da fatti eccezionali, infatti fino ad oggi così è stato, ma erano manifestazioni di un giorno che potevano comportare in qualche modo problemi di ordine pubblico. La seconda criticità riguarda la mancanza di una normativa comune sull'asilo. Questo è già stato detto, e lo ripeto: il primo, vero paradosso è che l'asilo si può chiedere solo se si arriva nel Paese nel quale presentare la domanda d'asilo, quindi il rifugiato deve arrivare sulle coste italiane o negli aeroporti italiani. E come ci arriva? Ci arriva con delle imbarcazioni clandestine? Così è stato fino ad oggi, quindi il problema è come poter permettere la presentazione di domanda d'asilo al di fuori dell'area di Schengen, quindi dell'area europea. C'è la proposta, ad esempio, di porre dei presidi in territorio libico, oggi garantiti dalla "*Coalition of the Willing*" o dall'Unione europea o da altre istituzioni internazionali. Questa potrebbe essere una via: presidi nei quali si possa fare domanda di asilo senza affrontare il rischiosissimo viaggio attraverso il Mediterraneo, che già ha causato centinaia, se non migliaia di morti negli ultimi quattro mesi. Questo è il

domani potrebbe essere qualsiasi altro Paese dell'Est Europa: se scoppiasse un Paese europeo o non europeo e ci fossero problemi, i rifugiati affluirebbero in Polonia, in Repubblica ceca, in Ungheria. ovvio che questo paradosso che oggi ci riguarda va in qualche modo sanato. Il terzo paradosso è quello della condivisione, che oggi è solo volontaria, la cosiddetta condivisione dell'onere. Filippi, per il sostegno di questi profughi? Tutti noi vorremmo una condivisione, vorremmo riconsegnare all'Europa un briciolo di sovranità, ma noi ce la siamo voluta tenere tutta la sovranità e quindi nessuno vuole questa condivisione, nessuno (l'Italia in testa) ha voluto la condivisione. in testa) ha voluto la condivisione. Oggi sono 60.000 le persone che hanno richiesto asilo in Italia; l'Italia ha un ottavo del PIL dell'Europa e ha un ventisettesimo dei rifugiati in Europa; l'Italia ha 60.000 rifugiati, ma la Germania ne ha 650.000, la Francia 250.000. La cosiddetta condivisione, il lamento per cui «l'Europa ci lascia soli» va inserito in questo quadro, e lo stesso Berlusconi, nella lettera scritta a Sarkozy, riconosce che la Francia ha fatto molto più di noi per quanto riguarda l'asilo. È scritto

l'Unione europea è stata assente. Vi sono 11 accordi di riammissione che riguardano i Paesi dell'oriente europeo, più Hong Kong e Macao;

Quindi, possiamo bombardare, ma non possiamo portare soccorso umanitario con EUFOR. Si tratta di un paradosso, di una criticità grande come una casa di cui però nessuno parla. Il ministro Frattini, che è molto loquace ed è molto generoso nelle sue conferenze stampa e nelle sue interviste,

umanitario. Ogni tanto si fa qualcosa, ma non c'è la bandiera italiana sopra la guida del soccorso umanitario per la Libia.

vorrei sottolineare il fallimento della politica migratoria italiana. Al senatore Filippi dico che il ministro Maroni dovrebbe dimettersi come ministro dell'interno.

Cito anche l'esempio della cosiddetta emergenza tunisina. Si sono tenuti 6.000 tunisini accatastati nell'isola di Lampedusa quando si potevano benissimo evacuare nel giro di 24 ore, come poi si è dimostrato, per farne uno spauracchio per l'Europa. Lo spauracchio era Lampedusa:

per rientrare dal debito e far crescere l'economia, occorrerà un quarto di milione di immigrazione netta nel nostro Paese. Vogliamo prendere o meno sul serio il tema migratorio e attuare una nuova

una politica europea, è stata completamente disattesa dagli incontri e dalle scadenze successive. È evidente allora ‑ concordo con il senatore Cabras ‑ che l'altro paletto non può che essere il Consiglio europeo che si riunirà dedicato proprio al tema al quale si sono riferiti i senatori Alberto Filippi e Livi Bacci. Ho l'impressione che, nella disattenzione europea di tutti questi anni,

Perduca ha notato come, in materia di dissidenti, che esistono e ne esistevano, nelle atroci prigioni - per esempio la disattenzione e l'inaffidabilità europea abbiano rasentato il cinismo, o peggio ancora. Da questo punto di vista, mi permetterei di utilizzare e di spostare,

prima e dopo, quando era più facile, la caduta del Muro di Berlino. Anzi, lo dico con un certo orgoglio europeo e italiano. Ricordo come una delle maggiori benemerenze del nostro Paese quella conferenza che l'onorevole Craxi volle si svolgesse a Venezia pochi mesi prima delle decisioni dei Paesi europei in materia di riarmo. Il Paese fu allora molto diviso; ci furono pressioni da parte del senatore a vita Agnelli e, addirittura, da parte del senatore Andreotti per limitare il visto di ingresso a Sacharov. Ci furono pressioni addirittura affinché non si rompesse con l'Unione Sovietica neanche nel momento in cui, proprio in quelle settimane, la segretaria di Solzenicyn veniva sottoposta a tortura. Ripensando a questa vicenda, non c'è dubbio che la nostra complessiva disattenzione ai dissidenti di quel mondo è stata colpevole, e aveva tutte le ragioni il collega Perduca nell'inserirla tra le questioni sulle quali l'Europa deve voltare pagina. pagina. A questo proposito, quando si dice che in tutti questi anni c'è stata una certa retorica nel concentrare l'attenzione sul conflitto israelo-palestinese e c'è stata nello stesso tempo, da qualche settimana, una insulsa retorica sulle cosiddette primavere di democrazia e di libertà dell'Islam, dobbiamo fare molta attenzione. In un passaggio del suo intervento, il collega Cabras attribuisce a un Paese europeo che pure dall'Europa non ha ricevuto

Non ho argomenti per contraddirlo, però non posso non ricordare la disattenzione e addirittura l'ostilità con le quali l'Europa ha voluto imballarsi in un ping-pong eterno nei confronti della Turchia, quasi a rimproverare a quel Paese le sue benemerenze di leale alleato dell'Europa e degli Stati Uniti nell'Alleanza atlantica.

la Turchia ha bussato all'Europa, gli Stati Uniti hanno chiesto all'Europa di aprirle le porte. Ovviamente, gli Stati Uniti erano interessati al rapporto con la Turchia ai tempi della guerra con l'Iraq. Mi pare che il Presidente del Consiglio italiano sia lo stesso di allora: lo si attaccò da parte dell'allora presidente della Commissione europea, il professor Prodi, per essere andato a un matrimonio estivo di un figlio di Erdogan, così come lo attaccarono allora Chirac e Schroeder. L'argomento

dell'accelerazione del rapporto con questo Paese. Quale che sia, non ho cognizioni tali per potermi pronunciare nello stesso modo del senatore Cabras sulla sua primavera di democrazia e di libertà civili, ma ho constatato però - lo abbiamo constatato in molti - che sullo scenario internazionale la Turchia, la Turchia, sentitasi respinta dall'Europa, ha guardato dall'altra parte, sempre meno a Occidente e in verso i Paesi del fondamentalismo islamico più aspro: la Siria e l'Iran. È un argomento del quale abbiamo parlato a lungo l'anno scorso, ai tempi della Flotilla e della nave Marmara. Ricordo con orgoglio di europeo e di italiano la prontezza e il coraggio delle valutazioni che proprio l'onorevole Sottosegretario fece quella mattina. Allora, da questo punto di vista, un anno dopo, c'è un'altra preoccupazione: non solo che la Turchia sia irrimediabilmente smarrita come alleato e interlocutore dell'Occidente, perché guarda verso altri orizzonti che cambierebbero la sua storia politica. In quella storia politica, intrecciata a livello diplomatico e di servizi di sicurezza con lo Stato israeliano, si parla oggi di una Flotilla 2, e con grande irresponsabilità si dice che vogliano partire dall'Italia e da altri Paesi europei. Si sono presentati, fortunatamente

l'argomento umanitario è vero e serio: non lo si può far diventare flaccido, come tante volte avviene. Ammesso e non concesso che ci fosse una Flotilla di 20 navi,

l'Italia deve svolgere il proprio ruolo, e bene ha fatto il nostro Presidente del Consiglio un mese e mezzo fa a dire alla radio israeliana che l'Italia avrebbe fatto tutto il possibile per impedire questa sciagurata partenza, che sarebbe un atto di retorica dell'ostilità ad Israele e della simpatia pregiudiziale verso Hamas.

In tutti questi anni si è parlato con molta retorica e con molti luoghi comuni di attenzione al Mediterraneo. L'ultimo dei fallimenti, ricordato dal senatore Livi Bacci, è stato il velleitarismo con il quale si è guardato all'Unione per il Mediterraneo. A questo proposito, mi sento di fare un'ultima considerazione: è mai possibile che con questi Paesi manchi del tutto una diplomazia dei Parlamenti? Non c'è riuscita l'Unione per il Mediterraneo: all'OSCE, dove il collega Livi Bacci è stato molte volte al mio fianco, ci sono cinque Paesi osservatori

l'aspetto della diplomazia parlamentare e fra Parlamenti non è affatto marginale. Sulla base di queste considerazioni, ritengo che il Senato abbia fatto bene, ieri e oggi, a discutere e ad approfondire

all'inizio del dibattito a proposito della definizione di diritti dell'uomo e non di diritti umani: è scritto nella risoluzione, ma credo che possiamo tranquillamente correggerlo. Non si tratta di un ritorno a prima degli anni Sessanta. Parto proprio da questa considerazione per riprendere un tema richiamato anche negli interventi di stamattina: quello del rapporto con i dissidenti.

praticata nel corso degli anni, non è più una linea che possiamo sostenere, in questo concetto si ricomprende anche il tema degli errori commessi nel rapporto con la dissidenza. Ovviamente, i due pesi e le due misure, diplomaticamente governati nel corso degli anni, sono ancora presenti nella diplomazia internazionale. Il primo esempio che mi viene in mente è il rapporto del mondo occidentale con la Cina, Paese che da questo punto di vista deve sicuramente guadagnare terreno sul tema dei diritti umani e delle libertà. Per essere coerenti con questa affermazione non vale mettere su un piatto della bilancia il peso degli scambi commerciali con la Cina,

il tema della politica migratoria, completamente assente nella sostanza concreta anche negli ultimi provvedimenti che la Commissione europea ha adottato, per esempio nella risposta - l'ho detto di integrazione alla relazione - alla lettera congiunta del presidente Berlusconi e del presidente Sarkozy. Quella risposta della Commissione è una sorta di riconoscimento della propria, almeno finora, incapacità ad essere adeguati ai problemi che la realtà sta proponendo. Ovviamente, noi confidiamo che anche questa discussione, questa risoluzione, la posizione che il Governo terrà nel Consiglio europeo del 24 giugno, il sostegno che noi vogliamo dare alla posizione del Governo in questa direzione, direzione, possano aiutare in un cambiamento profondo, e soprattutto nell'effettivo utilizzo dei nuovi strumenti che il Trattato di Lisbona consente, e che finora, come abbiamo ricordato, sono stati utilizzati in maniera non appropriata.

Dobbiamo, però, riconoscere che in quella vasta regione vi è un ruolo di *leadership* che sta entrando in discussione profonda, e che comprende il ruolo della Turchia e quello dell'Iran. Noi dobbiamo decidere quale atteggiamento assumere nei confronti della Turchia. Se la Turchia non può essere definitivamente un interlocutore a pieno titolo dell'Europa, e quindi dell'Occidente, giocoforza, per *realpolitik*, tenterà di essere *leader* dell'altra area, sganciandosi sempre di più dal rapporto che ha avuto finora con l'Occidente. Questo è il tema che dovrà svilupparsi nei prossimi tempi, e che anche

gli errori che stiamo probabilmente commettendo. Non credo che questo tema del negoziato, dell'ingresso della Turchia nell'Unione europea, possa essere ancora lasciato nella condizione nella quale si trova. Occorre prendere una decisione definitiva, perché questo può essere, effettivamente, l'elemento che fa pendere l'opinione politica e, soprattutto, il ruolo di quel Paese in una direzione piuttosto che in un'altra. Posso sbagliare, ma credo che questa sia una delle questioni sulle quali nei prossimi mesi dovremo ulteriormente tornare. *(Applausi dal Gruppo

pone l'Europa in attenzione verso il Mediterraneo circa 14 anni fa. Quindi, da un certo punto di vista, non si può neppure dire che l'Europa non abbia avvertito nel tempo una sensibilità particolare per il Mediterraneo. Vorrei aggiungere che, evidentemente, in questo ultimo decennio qualcosa è cambiato in Europa, perché, tanto per ricordare una vicenda che oggi torna attuale, durante la Presidenza italiana dell'Unione europea, e anche durante la Presidenza spagnola, che precedeva precedeva la nostra e con cui eravamo in rapporto, fu chiesto di istituire una banca di finanziamento, legata al Processo di Barcellona, per quanto riguardava le questioni dello sviluppo nel Mediterraneo.

E ciò dimostra che, forse, la disattenzione dell'Europa verso il Sud del Mediterraneo nell'ultimo periodo è aumentata. Si dice che il Processo di Barcellona è fallito: ci sono ovviamente delle responsabilità europee,

Voglio ricordare, per esempio, che così come giustamente ci lamentiamo del fatto che i rapporti commerciali tra Nord e Sud del Mediterraneo siano molto bassi rispetto al potenziale, forse bisognerebbe anche osservare che i rapporti Sud‑Sud sono ancora più bassi dei rapporti Nord‑Sud, e cioè che esistono problemi insiti e strutturali anche all'interno dell'area nordafricana.

Vogliamo ricordare il popolo Saharawi, la chiusura delle frontiere tra Marocco e Algeria, i motivi per cui non è decollato il Maghreb e il cosiddetto «5+5» non ha funzionato, ma se non ci rendiamo conto di questi passaggi o di questi blocchi, che la storia e la cronaca hanno consentito, oggi

anni fa, da un Presidente della Repubblica, che può piacere o non piacere, ma che comunque è a capo di uno dei più importanti Stati europei, ed ebbe una grande risonanza, perché furono invitati alle celebrazioni dell'indipendenza francese i maggiori esponenti e i Capi di Stato di quest'area),

allora che qui sia stato fatto un grosso lavoro, proprio perché si è lavorato nell'ottica giusta, europea, quella che valuta ciò che è possibile nel contesto nel quale operiamo. c'è anche, credo, l'unanimità da parte delle forze politiche, anche se poi nel dibattito si è visto che, sotto sotto, come è chiaro, restano alcune profonde differenze e alcune insoddisfazioni. Ma, al di là di questa, che è una linea di indirizzo che il Parlamento dà al Governo anche per rafforzare la posizione dell'Esecutivo all'interno di un dibattito europeo, vorrei ricordare timidamente che tale dibattito è sempre meno simile a quello immaginato a Lisbona e sempre più simile a quello che c'era prima

perché resta ancora un'impostazione - è sotto gli occhi di tutti - molto più simile all'Europa intergovernativa che non a quella comunitaria per la quale molti di noi avevano lavorato e sperato, e tutt'ora lavorano e sperano. prendiamo questa risoluzione nella sua valenza, nella sua importanza politica, direi anche nella sua capacità politica di aver impegnato non solo la Commissione, ma l'Aula, come giustamente si è voluto, per dare anche una certa risonanza,

Credo che tutti noi stiamo faticosamente cercando la strada verso l'integrazione in un mondo che sta profondamente cambiando.

lo vado dicendo da una vita, e sono oramai stanco di ripeterlo: il problema sono le tragedie degli ultimi giorni, sono gli ultimi immigrati, sono i disperati della Terra, è il mezzo milione di africani del Sub-Sahara che era in Libia e che è solo l'avanguardia

è anche questo. Infatti, mentre per la politica di vicinato del partenariato orientale abbiamo trovato 600 milioni di euro, non abbiamo trovato neppure un decimo di tale cifra per l'Unione per il Mediterraneo e per il Processo di Barcellona. Questo è un dato di fatto

a qualcuno aveva anche lanciato il segnale del fatto che questo pilastro egiziano non era poi più così forte in prospettiva. Certamente si sono combinati poi due fattori: una nuova politica turca più attenta al vicino, ma nello stesso tempo anche la necessità di avere qualche altro punto di riferimento nell'area del Mediterraneo orientale, che potesse in qualche modo garantire o sopperire ad alcune debolezze.

allora sono stati anche quelli di non avere forse forzato gli strumenti che avevamo, di democrazia parlamentare, per esempio, per far cambiare a questi Paesi quello che era solo un disegno teorico. Ricordo di essere stato al Parlamento algerino, al Parlamento tunisino, a quello egiziano, e di aver accompagnato Presidenti della Repubblica italiana che venivano invitati dai Presidenti evidentemente, ci siamo limitati all'aspetto formale, nel senso che abbiamo visto delle persone attorno a un emiciclo, pensando che fosse democrazia, e forse dovevamo invece operare con maggior attenzione, o forse anche valorizzare gli strumenti che avevamo per avvertire

di dover dire al Parlamento che esistono altre motivazioni per trovare occasioni dove approfondire un dibattito che deve portare l'Europa a cambiare, non dico politica, ma l'approccio, la cultura dell'Europa verso il Mediterraneo, ricordando che non è una frontiera della paura - come molte volte si avverte - ma è la frontiera nella quale dobbiamo misurarci tutti i giorni e nella quale comunque noi siamo inseriti.

e mi permetto solo di segnalare che in alcune Istituzioni si comincia a parlare di «diritti della persona»: lo sottolineo perché mi sembra una formula più adeguata da molti punti di vista; è poi l'Aula che sceglie, ma

critica forte sia politica, sia sugli strumenti per risolvere questa crisi, e sugli strumenti finanziari carenti che sono stati fino ad oggi previsti. È una risoluzione importante, perché dà utili consigli all'Unione europea per proseguire in maniera diversa nei rapporti con la sponda Sud del Mediterraneo, per dare maggiori istruzioni e coesione ai Paesi membri per affrontare un problema fondamentale come quello dell'immigrazione e dei profughi che vengono dal

Purtroppo, ritenendo importante che l'Assemblea del Senato discuta di questo provvedimento, sono rammaricata dal fatto che la stessa Assemblea decida di occuparsene da un giorno all'altro, quando molti dei senatori che siedono in Commissione esteri sono impegnati in missione. Fatta questa doverosa premessa - doverosa, colleghi, perché credo che vista la portata dei temi trattati sarebbe stato opportuno occuparsene con cognizione di causa e non per riempire la scaletta del calendario dei lavori - mi accingo ad esprimere il voto favorevole del mio Gruppo sul testo che oggi votiamo. Vorrei, però, aggiungere qualche piccola considerazione. L'Italia dei Valori ritiene che la scelta operata dalla Commissione europea e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri di predisporre prima una comunicazione congiunta, cui far seguire un rinnovato partenariato a sostegno del cambiamento in tutto il Mediterraneo meridionale, sia stata una scelta giudiziosa. Noi dell'Italia dei Valori, anche e soprattutto in conseguenza dei gravi e numerosi accadimenti occorsi negli ultimi due-tre anni - mi riferisco agli sbarchi di migranti (non "clandestini", come qualcuno preferisce chiamarli), alla diminuzione della ricchezza *pro capite* nei Paesi del Nord Africa, all'acuirsi delle condotte dittatoriali o paramilitari che hanno preceduto di gran lunga le crisi scoppiate negli ultimi mesi - avevamo già fatto delle proposte. Non è la prima volta che si discute di questi problemi in quest'Aula in questa legislatura. Ne abbiamo parlato, infatti, ogni qualvolta l'agenda del Governo, dettata dalla Lega Nord, riportava all'ordine del giorno pacchetti sicurezza, trattati con dittatori o atti simili. Spesso abbiamo chiesto al Governo di avere un atteggiamento diverso nelle relazioni internazionali con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e di perseguire un altro tipo di politica comunitaria. L'obiettivo - che da sempre abbiamo considerato di importanza strategica - di un rinnovamento delle relazioni dell'Unione con i propri vicini meridionali è sicuramente opportuno, perché è interesse comune che il Mediterraneo meridionale sia una zona democratica, stabile, prospera e pacifica. Un nuovo partenariato è quindi di fondamentale importanza, ed è ancora più importante che questo nuovo partenariato realizzi gli obiettivi che le istanze che ho richiamato si prefiggono. Come leggo dall'atto comunitario n. 71, la UE «intende mettere a disposizione dei Paesi del Sud del Mediterraneo, che abbiano la capacità e la volontà di avviare le trasformazioni necessarie per un cammino verso lo Stato di diritto, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti umani e il pluralismo, le proprie competenze a tutti i livelli e con un'impostazione differenziata, secondo la specificità di ogni situazione». Per fare ciò, sono state previste delle misure urgenti, tra le quali uno stanziamento di 30 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere nell'immediato la popolazione libica e le popolazioni sfollate presso le frontiere tunisine ed egiziane; un'agevolazione della cooperazione consolare e dell'evacuazione; il ricorso ai 25 milioni di euro del Fondo UE per le frontiere esterne e del Fondo europeo per i rifugiati; strumenti per sostenere l'Italia, e se necessario altri Stati membri, nell'eventualità di un arrivo in massa di migranti dall'Africa settentrionale; stanziamento di 17 milioni di euro per l'assistenza alla Tunisia, sia come sostegno alla società civile, sia in termini di assistenza per la transizione verso la democrazia e verso le elezioni; misure restrittive verso il regime libico, compreso il congelamento dei capitali. Per il medio-lungo periodo apprendiamo dal testo che «la Comunicazione congiunta indica invece come assoluta priorità la ridefinizione delle politiche UE nei confronti dei suoi *partner*». In particolare si ritiene che la nuova impostazione debba basarsi sugli incentivi, sul concetto di *more for more*, vale a dire maggiori aiuti per quei Paesi che più velocemente portano avanti le necessarie riforme e, viceversa, cancellazione degli aiuti per coloro che non rispettano o abbandonano i piani di riforma concordati. Faranno parte dei piani di riforma anche le questioni di genere, che svolgeranno un ruolo chiave per il futuro sostegno UE. Il requisito fondamentale per poter accedere al partenariato è l'impegno per elezioni libere ed eque ma anche per un lavoro congiunto nelle sedi internazionali su questioni di interesse comune. Si presuppone quindi un dialogo politico più intenso rispetto al passato. Il partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa, oltre che seguire il principio del *more for more*, dovrà incardinarsi su tre elementi: trasformazione democratica e sviluppo istituzionale con particolare attenzione alle libertà fondamentali; rapporto più forte con la popolazione e sostegno alla società civile; crescita e sviluppo economico sostenibili e inclusivi. L'Italia dei Valori condivide pienamente gli intenti contenuti nel documento che stiamo trattando, ma è ancor più favorevole nei confronti degli importanti impegni ai quali il Governo è richiamato dal testo della risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione. Ricordo solo alcuni di questi, colleghi, «a destinare ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo risorse della politica di vicinato, adeguate al perseguimento degli obiettivi esposti»; «a perseguire l'obiettivo di dare maggiore visibilità all'azione dell'Unione europea attraverso forme di sostegno all'economia locale, allo sviluppo di infrastrutture nonché al rafforzamento delle istituzioni»; «a garantire il massimo coordinamento tra tutte le politiche dell'Unione»; «a promuovere una effettiva politica comune in materia migratoria e di gestione delle frontiere in ambito UE e l'istituzione, entro il 2012, di un Sistema comune europeo d'asilo al fine di garantire quell'essenziale principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri previsto dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; a coordinare «in particolare le politiche di assistenza umanitaria, cooperazione allo sviluppo». Questi sono gli impegni che ci interessa raggiungere in una nuova Europa, e siccome l'Europa altro non è che la somma di tanti Governi nazionali, noi dell'Italia dei Valori ribadiamo l'invito al Governo a battersi nelle sedi opportune affinché anche gli altri Stati europei si spendano in tale direzione, e pertanto votiamo favorevolmente. Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, quasi sei mesi ormai di rivoluzioni, in parte compiute, in parte ancora drammaticamente in corso, segnano una svolta epocale anche per l'Europa e per il mondo, al pari della fine del colonialismo o della caduta del Muro di Berlino. Ci sono molte cause, di cui abbiamo parlato molte volte - la crescita demografica assai rapida, la scolarizzazione,

che tuttora talora sussistono o stanno cadendo, determinando negli anni un clima di diffusa ingiustizia sociale. Questa pressione ha determinato la spinta alla modernizzazione, alla democratizzazione che oggi abbiamo sotto i nostri occhi. Sono spesso stati sottovalutati - vorrei ricordarlo - gli aspetti economici di questa dinamica. A fronte di una crescita della popolazione molto importante, dell'ordine del 30 per cento negli anni 2000, contro una crescita zero dei dirimpettai europei, il PIL *pro capite* è cresciuto di oltre di oltre il 100 per cento in media nei Paesi del Nord Africa. Il commercio estero è cresciuto da un minimo del 146 per cento della Tunisia a un massimo del 380 per cento dell'Algeria; è stata sottovalutata anche la crescita dei rapporti con l'Italia: l'interscambio con l'Italia, prima della crisi economica, era arrivato a 27 miliardi di euro, ovverosia più del doppio di cinque anni prima e più del triplo di 10 anni prima. Si è determinata una sorta di trialismo mediterraneo tra l'Europa occidentale (crescita demografica ed economica molto contenuta, quando non zero), Europa orientale, balcanica e bacino del Mar Nero (crescita demografica molto contenuta o zero, ma crescita economica importante) e Mediterraneo meridionale, caratterizzato da queste dinamiche di crescita molto forte. la geopolitica del bacino del Mediterraneo: fin qui c'è stata, se vogliamo, una crescita pur in assenza di democrazia, ma questa democrazia che sta arrivando in questi Paesi ci lascia pensare che produrrà ulteriore crescita. Il rapporto fra democrazia e crescita economica è controverso: Amartya Sen teorizza che sia rigorosamente positivo; alcune evidenze, soprattutto del Sud-Est asiatico, ci suggeriscono un'altra cosa; ma nei Paesi di cui parliamo oggi probabilmente sarà ulteriormente positivo, perché

aumenterà la concorrenza all'Europa da parte loro e aumenterà la concorrenza all'Europa da parte di altri Paesi per penetrare su quei mercati che una volta erano principalmente appannaggio dei loro dirimpettai, e cioè dei Paesi del Sud Europa. Questa è una considerazione aggiuntiva rispetto alle giuste preoccupazioni per l'instabilità e per i possibili conflitti, le possibili derive oltranziste e confessionali che si annidano in questa impetuosa dinamica. Naturalmente, se questo è il contesto (ed è più o meno questo, anche se l'ho imperfettamente riassunto) pesa più che mai - è stato ricordato da tutti - l'assenza di una strategia dell'Unione europea per il Mediterraneo. Il fallimento del Processo di Barcellona e dell'Unione per il Mediterraneo avviene sostanzialmente perché essi si basavano sul presupposto di continuare a sostenere i regimi esistenti: nella migliore o più benevola delle ipotesi, per evitare delle derive oltranziste; nella forse meno benevola delle ipotesi, per non spartire con quei Paesi i benefici della loro crescita. Non dimentichiamo che, anche se il PIL *pro capite* in

tassi di crescita. Ebbene, rispetto a tutto questo, il senso di questa risoluzione, che è proprio intitolata alla democrazia e alla prosperità condivisa, mi pare assolutamente evidente. Mi pare assolutamente evidente e giusto che quest'Aula cerchi di indicare la direzione di una nuova politica mediterranea per l'Europa, in cui l'Italia, per il proprio ruolo storico e geografico, torni a svolgere una funzione trainante. sostanzialmente condivisibili tutte le istanze in essa richiamate, in particolare nella parte impegnativa, salvo forse ritenere che possano essere qua e là un po' ingenue, o che possano comunque difficilmente produrre gli effetti, che talora addirittura sono già scritti, ma che semplicemente non si producono per la mancanza di una volontà politica in questo senso. promuovere la politica comune in materia di migrazioni e di gestione unitaria delle frontiere esterne, peraltro già radicata nell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come mi pare abbia ricordato il senatore Alberto Filippi. d'accordo su una nuova politica di vicinato che incentivi l'accettazione e la promozione di principi democratici e diritti umani e civili, e concordo anche sul sostegno politico agli interventi della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca europea per gli investimenti condizionati a riforme economiche; ma attenzione, perché su quello scenario sempre gioco più facile i *donors* o gli investitori che non chiedono niente in cambio, rispetto a quelli che chiedono riforme civili e, se posso dire, anche rispetto alle astruse procedure che talvolta i progetti europei prevedono. Forse, quindi, si poteva e si doveva usare qualcosa di un un po' diverso rispetto alla cooperazione economica, pensare più a una crescita complementare tra le regioni sulle due sponde del Mediterraneo, una crescita dal basso, applicare le strategie di reti di imprese e reti di sistemi economici territoriali, puntare sulla complementarietà tra i fattori produttivi, anche attraverso una politica delle migrazioni che miri ad una selezione quantitativa e qualitativa. Qualcuno ha detto che le frecce dei migranti dicono dove va la storia: ebbene, le frecce dei migranti ci trapassano dolorosamente e vanno da un'altra parte, e la storia pure. Questo sta succedendo: noi siamo terra di nessuno non solo per l'Unione europea, ma siamo purtroppo terra di nessuno anche per i migranti, che passano di qui perché è più comodo, ma quasi sempre vogliono andare da un'altra parte.

- avrà effetti anche sull'Europa dal punto di vista del migliore utilizzo dei fattori produttivi, anche europei, della maggiore possibilità di penetrare o restare su mercati certamente in crescita, come quelli di cui stiamo parlando, e di un rallentamento e di una migliore qualificazione dei flussi migratori. Il solo rischio - lo affermo in conclusione, preannunciando il voto

è sbagliata. Quest'Assemblea dovrebbe smettere di pensare che gli argomenti europei debbano essere inseriti e calendarizzati in Aula come riempitivo quando non si sa cosa fare di meglio, oppure per dimostrare che comunque il Senato lavora qualche ora in più.

Innanzitutto, la risoluzione tratta quella che dovrebbe essere la politica estera dell'Unione europea; la migrazione rappresenta soltanto una parte della politica estera dell'Unione europea, ma qui si vanno a toccare temi molto importanti. Concordo su tutti i punti sollevati,

il partenariato orientale che ha portato via fondi e risorse a quella che era la politica mediterranea. Quanto ai fondi,

trovare fondi per questa importante politica che noi dovremmo fare nei Paesi dell'Africa, e in

Tunisia, FRONTEX - e dell'implementazione di tali meccanismi. Pertanto, non è vero che siamo tornati a casa con le cosiddette pive nel sacco e non abbiamo ottenuto assolutamente nulla.

cercare di coinvolgere questi Paesi almeno come uditori al Consiglio d'Europa, perché la reputo un'idea valida. Ancora, credo vada assolutamente supportata la richiesta che la Commissione chiarisca bene, a proposito della direttiva n. quali sono gli effettivi momenti in cui si registra un flusso particolarmente forte di migranti.

anche per il nostro Gruppo dai colleghi intervenuti nel corso della discussione. Il primo giudizio riguarda quanto sta avvenendo nel Mediterraneo. Siamo in presenza di una svolta storica una svolta storica che chiude una fase; una fase nella quale sembrava impossibile uscire da un'alternativa perversa: una parte, un Islam fondamentalista, che usava la religione islamica come ideologia totalitaria, in una sorta di via arabo‑islamica alla nazionalizzazione delle masse, conosciuta dall'Europa nel Novecento con altri totalitarismi; dall'altra parte, come unica alternativa, regimi eredi anche di storie non banali e non ignobili (pensiamo alla storia dell'Egitto o a quella, come ricordava il sottosegretario Mantica, della Tunisia e dell'Algeria: i partiti nazionali della decolonizzazione, della lotta per l'indipendenza e per la libertà, che avevano costruito regimi nazionalisti e autoritari), che però sono diventati regimi di polizia tendenzialmente corrotti. L'alternativa per l'Europa e per l'Occidente sembrava essere chiusa in questa difficoltà. La Presidenza Bush, per la verità, ha tentato un'uscita da questa alternativa con l'avventura irachena,

Sappiamo come è andata a finire: quell'avventura ha prodotto disastri da ogni punto di vista: anzitutto, dal lato del rapporto col mondo arabo-islamico, per non parlare delle centinaia di migliaia di vittime e del rafforzamento dell'Iran, che è stato l'unico vero beneficiario di quella avventura bellica. Tuttavia, il problema rimaneva, centrale. A quanto pare, si stanno decidendo a risolverlo, o perlomeno ad affrontarlo in maniera determinata, i popoli della sponda Sud del Mediterraneo, del Medio Oriente e del Golfo, in un processo del quale è impossibile non cogliere tutti i rischi, le tensioni e le difficoltà, ma del quale tuttavia dobbiamo cogliere anche la straordinaria opportunità. In sostanza, cosa c'è alla base di quello che il Presidente della Repubblica ha chiamato il Risorgimento arabo (mentre comunemente è definito come la "primavera araba")?

il pensiero prevalente nel modo arabo islamico era che la globalizzazione fosse una sorta di americanizzazione forzata del mondo, che avrebbe costretto il mondo arabo-islamico stesso ad una persistente condizione di subalternità. Oggi, l'analisi sulla globalizzazione è radicalmente cambiata: è invalsa la definizione di successo di quello

E allora i giovani - quella metà della popolazione del mondo arabo-islamico che ha meno di 25 anni e che in gran parte è una generazione istruita cominciato a ragionare su questo e a chiedersi: perché noi no? Perché noi non possiamo essere, come gli altri, protagonisti della globalizzazione? Se non lo siamo, non è tanto o solo colpa dell'America cattiva o dell'Europa dell'Europa tardo-coloniale, ma la responsabilità prima è nostra, e la causa va innanzitutto trovata qui. Sono questi regimi, è il sistema statuale, politico e politico-economico dei nostri Paesi che non funzionano e che non sono all'altezza, né in grado di portarci in modo efficace dentro la globalizzazione.

gli Stati Uniti si sono fatti forza della discussione che aveva avuto luogo nell'era Bush: tutti sanno come fossimo certamente e chiaramente dall'altra parte, ma non si può non riconoscere ai neoconservatori quest'intuizione, e cioè che il problema della democrazia nel mondo arabo era cruciale e centrale. Tuttavia non è stato ancora risolto, anche se è stato affrontato in maniera determinata, ed è uno dei punti cardine della

Certo, un conto sono le intenzioni politiche generali e altra cosa è trasformarle in politica quotidiana. Sappiamo quanti siano le contraddizioni e i problemi; tuttavia, gli Stati Uniti hanno scelto chiaramente un indirizzo,

uno dei grandi europeisti, uno degli euro-entusiasti d'Italia, ha dovuto dire che l'Europa si è mossa in modo deludente su questa vicenda e quindi serve un salto di qualità dell'iniziativa europea.

meno intergovernativa. Tale questione non si può affrontare Paese per Paese, ognuno mosso soprattutto dalle ragioni miopi del proprio immediato tornaconto. Si può affrontare seriamente solo se l'Europa si muove come Europa; certo, trainata dai Paesi della sponda Nord del Mediterraneo, del fianco Sud dell'Europa. Se non sono loro, e l'Italia *in primis*, a cercare di spostare questo baricentro, chi ci aspettiamo lo faccia? La Danimarca, la Svezia, l'Estonia? È evidente che deve essere l'Italia. Questo è il terzo punto del mio ragionamento: il nostro interesse nazionale è avere un Mediterraneo che diventi una grande area di pace e di sviluppo nel mondo. E lo può diventare, oggi c'è l'occasione storica perché lo diventi. Allora, qual è il nostro interesse nazionale, se non questo? Pensiamo soltanto al tema del Mezzogiorno. Quale strada c'è per il Mezzogiorno d'Italia se non scommettere su un

ce lo dice l'articolo 11 della Costituzione - ci vuole coraggio e lungimiranza. L'articolo 11 della Costituzione ci dice che l'Italia deve promuovere un ordine internazionale fondato sulla giustizia e sulla pace attraverso limitazioni di sovranità. È tutto È tutto scritto: dobbiamo scommettere sulla primavera arabo-islamica, e dobbiamo farlo facendo crescere l'Europa , cioè con più Europa, a cominciare - e qui concludo - dal governo dei flussi migratori. Questa è la grande sfida del nostro futuro.

A Bruxelles si calcolano 20 milioni di nuovi immigrati di qui al 2050, cioè il raddoppio dell'attuale livello. Questa è una sfida gigantesca, della quale giustamente la senatrice Boldi ha messo in luce tutte le difficoltà e le criticità, che vanno affrontate con coraggio, come ha saputo fare il Parlamento europeo. La mozione Provera, ricordata dalla relazione del collega Cabras, indica una strada. Allora, smettiamo di fare cattiva propaganda su questo punto e cominciamo insieme a fare buona politica.

per dire che è un argomento che abbiamo già esaminato ampiamente sia in Commissione sia nelle informative che il Governo ha dato al Parlamento, Camera e Senato, in Aula e in Commissione. Per questo, vorrei cogliere l'occasione

nel mondo, hanno continuamente seguito e ascoltato il Parlamento. Ecco perché credo che - lo diceva il il documento che stiamo esaminando sia anche un promemoria - non dico un suggerimento, perché sarebbe troppo - un punto di riferimento

sono state anche messe in evidenza delle insufficienze nel regolare una situazione che è scoppiata all'improvviso, si è dilatata

È vero che l'interesse di singoli Paesi, fino adesso Francia e Germania in primo luogo, ha impedito una strategia dell'Unione europea in questo settore.

essere la regista delle economie di alcuni dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea. Se tutto questo è vero, il

del cambiamento in tutta la regione del Mediterraneo, è un nuovo partenariato, che però ha bisogno ancora di approfondimenti e di dilatazioni. Questo nuovo partenariato (e sottolineo il termine «nuovo», perché il vecchio lo abbiamo già, in qualche modo, indicato come insufficiente in queste situazioni)

comprende misure a breve termine, come lo stanziamento di circa 80 milioni di euro per un'azione di aiuti

Paesi. Questo nuovo partenariato va completato con quanto noi abbiamo chiesto e che figura nella risoluzione che stiamo esaminando. In particolare, i due aspetti di cui parlava ieri mi appaiono particolarmente importanti: le iniziative multilaterali e, soprattutto, il riferimento ai nuovi strumenti proposti e portati avanti dal Trattato di Lisbona. Signora Presidente, facendo salva l'analisi che abbiamo fatto, prendendo come punto di riferimento quanto Parlamento europeo, Consiglio e Commissione ci propongono, ma completato con le obiezioni, le